salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato», del quale iniziamo l'esame in Aula, costituisce un momento particolarmente significativo nel procedimento di riorganizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato iniziato sin dagli anni Novanta con le prime misure adottate dai Governi di allora. L'originaria proposta di riordino dei Dicasteri prevedeva di istituire il Ministero della sanità e delle politiche sociali, da un lato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'altro; tale progetto rimase inattuato a causa della crisi del Governo Ciampi. Fu invece con l'attuazione della delega conferita dalla cosiddetta legge Bassanini 1, che - nell'ambito di una riforma dell'organizzazione del Governo intesa a razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri, anche attraverso interventi di riordino, soppressione e fusione - si previde l'istituzione di un unitario Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il decreto legislativo n. 300 del 1999, che così disponeva individuando i 12 Dicasteri in cui si sarebbe articolata la struttura del Governo, non ha peraltro avuto attuazione sul punto fino al 2008: il nuovo assetto dell'Amministrazione centrale - applicabile a partire dalla XIV legislatura - fu modificato prima ancora di entrare in vigore, ad opera del decreto-legge n. 217 che portò a quattordici il numero dei Ministeri, re-istituendo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero della salute (già della sanità). Anche il successivo intervento in materia - posto in essere all'inizio della XV legislatura (in una fase sostanzialmente contestuale alla formazione del Governo)

È con la legge finanziaria 2008 che si torna a fissare in 12 il numero massimo di Ministeri, a partire dal Governo successivo a quello allora in carica, e cioè questo, senza peraltro individuarne né la denominazione né le competenze. Il nuovo assetto del Governo ha trovato attuazione all'inizio della legislatura in corso: il decreto-legge 16 giugno 2008, n. 85, ha infatti individuato i 12 Ministeri e ha disciplinato il trasferimento delle competenze e delle risorse umane,

accanto alla nomina del Ministro senza portafoglio per il turismo e all'attribuzione del titolo di Vice Ministro a cinque Sottosegretari, è stato approvato il disegno di legge ora all'esame dell'Assemblea. Nel rinviare alla relazione scritta per quanto riguarda la puntuale analisi del provvedimento, desidero ricordare che nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali anche i rappresentanti dell'opposizione hanno espresso il loro avviso favorevole all'istituzione

come è stato affermato correttamente dalla senatrice Adamo - un Ministero *ad hoc* in materia è in grado di rappresentare un ente di riferimento di grande utilità per l'interlocuzione con le Regioni. È questo il punto. Lo stesso senatore Bianco, in Commissione, ha evidenziato il fatto che non si può prescindere da una politica sanitaria unitaria a livello qualitativo, come testimonia l'azione del Governo, che si saldi con la competenza regionale che è garantita dall'articolo 117 della Costituzione e che deve vedere lo Stato e le Regioni lavorare in un processo di cooperazione e collaborazione istituzionale. la concentrazione di poteri, che pure è stata evidenziata da qualche intervento dell'opposizione su questo provvedimento, nelle mani del Ministero dell'economia deriva da un fatto che è sotto gli occhi di tutti: la spesa sanitaria rappresenta il volume di spesa più grande che è oggi nelle mani delle Regioni e spesso si determinano dei buchi di bilancio nei *budget* che le Regioni hanno a disposizione per coprire le esigenze della sanità. È quindi giusto che ci sia un processo di collegamento di collegamento costante e unitario con l'azione del Governo e un controllo che eviti poi procedure che portino al commissariamento nel settore della sanità, operando in prevenzione e facendo il collegamento unitario della politica della sanità non dopo che il danno è stato fatto, ma mentre la spesa va avanti.

il Governo venga a riferire annualmente in Parlamento, è una misura che può essere introdotta nel provvedimento proprio per sancire questo processo di cooperazione e collaborazione considerato che il Parlamento deve poi essere il destinatario finale delle informazioni per le decisioni che deve assumere. Con questo spirito cominciamo la discussione generale su un provvedimento che io credo meriti l'approvazione del Parlamento. *(Applausi

Signor Presidente, noi abbiamo posto una questione pregiudiziale di costituzionalità per tre ordini di ragioni. Una prima ragione riguarda la circostanza che, non per colpa nostra, la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha determinato un assetto e un sistema delle competenze in forza dei quali il Ministero per la salute, o della salute, era stato soppresso. Esso era stato soppresso perché, come è noto,

reintrodurre una struttura ministeriale e statale di controllo e di programmazione su tutto il territorio nazionale (non solo delle prestazioni minime e dei diritti fondamentali legati all'assistenza), ma riteniamo che il complesso dell'assistenza sanitaria e delle politiche di prevenzione debba essere essere e tornare totalmente in capo allo Stato sia perché vi sia una unica ed efficace *governance* in una materia così delicata e vicina ai bisogni degli cittadini sia perché, come dimostrato purtroppo dai fatti, l'ampliamento a dismisura della spesa pubblica sanitaria ha determinato un buco di bilancio non solo nelle Regioni del Sud ma anche in tante Regioni del Nord, non garantendo efficienza

peraltro non in linea con il dettato dell'articolo 117 della Costituzione; ci sembrerebbe - e ci sembra - più utile, onesto, chiaro e anche funzionale alla riorganizzazione di un Ministero che si occupi di questi problemi problemi la modifica dell'articolo 117 della Costituzione. Solo attraverso la modifica del sistema delle competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria si potrà, decisamente e realmente, garantire un sistema efficace di governo su questi problemi, soprattutto allorquando le Regioni non sono attrezzate, ad esempio, per fronteggiare in maniera omogenea ed efficace temi come quelli che in questi momenti viviamo. Mi riferisco alla nuova forma di influenza virale e ad altri nostra considerazione è sempre legata al dettato costituzionale, perché la prova provata che questo provvedimento è o inutile o in totale contrasto con la Costituzione lo dà proprio la legge delega sul federalismo fiscale che questa maggioranza ha approvato qualche mese fa. Tale provvedimento enuncia un principio in forza del quale ad ogni struttura amministrativa che si costituisca in capo allo Stato e alle Regioni in forza di competenze e funzioni amministrative assegnate deve corrispondere un taglio ed una soppressione di altra struttura che si occupi della stessa materia. Siamo qui in presenza di una sovrastruttura, cioè di una nuova struttura burocratica che si costituisce in capo allo Stato senza che si abbia peraltro certezza delle competenze

pregiudiziale - alla violazione dell'articolo 81 della Costituzione, non corrisponde una soppressione di uffici, di competenze, di personale e di risorse ad altri livelli territoriali di Governo a cui si ritiene si sottraggano queste competenze. Siamo in presenza dell'ennesimo provvedimento che testimonia la schizofrenia politica ed istituzionale di questo Governo e di questa maggioranza, che da un lato parlano di federalismo istituzionale e di decentramento di federalismo istituzionale e di decentramento e, dall'altro, con atto amministrativo reintroducono il Ministero del turismo, anch'esso oggetto sconosciuto e inutile

ha trasferito troppe competenze alle Regioni determinando il disastro della sanità in tante Regioni e l'ingovernabilità sotto il profilo della spesa pubblica di questo settore delicato. Queste sono alcune delle ragioni che ci hanno indotto a sottolineare

di mera consulenza e assistenza, di sovrintendenza ma senza alcun potere reale rispetto a ciò che le Regioni fanno nel campo sanitario sarebbe ancora più grave perché l'inutilità testimonierebbe, in questo momento particolare della finanza pubblica, la necessità di regolare meglio conti politici all'interno della maggioranza portando a 13 il numero dei Ministeri senza alcuna reale motivazione e senza nessuna reale

centrale della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione e, in particolar modo, della riforma dell'articolo 117 della Costituzione che tanti disastri,

finestra"). Ricordo che sulla questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si svolge un'unica discussione, durante la quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

sue argomentazioni giuridiche sono sempre estremamente pregevoli. Mi pare tuttavia che in questa occasione la posizione del suo Gruppo sia di bandiera, non facilmente comprensibile e non in linea con quanto è accaduto negli anni in relazione alla materia che stiamo trattando. Sono stato il relatore del provvedimento di ripacchettamento del giugno dell'anno scorso e ricordo perfettamente che furono presentati dalla maggioranza, ma anche dall'opposizione, diversi ordini del giorno, accolti dal Governo in quel momento, tesi a ristabilire il Ministero della salute. Non ricordo se ci fu anche un ordine del giorno dell'UDC-SVP-Aut, però l'opposizione così come la maggioranza, lo ripeto, si determinò in questo modo. La risposta del Governo fu quella di accogliere gli ordini del giorno e di vedere per il futuro come muoversi per la ricostituzione del Ministero della salute. Siamo arrivati a questo punto, come ha spiegato molto bene il relatore Vizzini. Quelle esigenze che già erano evidenti nel giugno 2008 si sono rese ulteriormente urgenti con tutta una serie di problemi che vedono il Ministero della salute al centro di tante materie, di tante operazioni, di tanta necessaria specificazione generale dei problemi, e siamo arrivati a questo provvedimento - oggi al suo

chiaramente alla competenza dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale mentre, in termini di competenza concorrente Stato-Regioni, è vero che la tutela della salute è attribuita alle Regioni, ma residua

corretta base per il provvedimento che voteremo. Sul fatto poi che ci sia da parte del senatore D'Alia la critica alla copertura, quindi la violazione dell'articolo 81, devo dire che questa impostazione è tenuta sul generico, senza precise indicazioni. che tutta la struttura del provvedimento, ivi comprese le coperture, e anche il ricorso all'operatività del Ministero dell'economia tendano a dare la precisa impressione - più che un'impressione è una realtà - che il disegno di legge sia costituzionale sul piano dei princìpi dell'articolo 117 e sia costituzionale sul piano dei princìpi dell'articolo 81, perché la copertura, l'impostazione e l'intervento del Ministro dell'economia tendono proprio a garantire un'ampia copertura economica. D'altro canto, come ricordava il presidente Vizzini, il Governo Prodi stabilì l'autonomia del Ministero della salute: quindi, vuol dire che già si era pensato e deciso concretamente di lasciare al Ministero della salute quelle competenze in vigenza già allora - parliamo del 2006 - della riforma costituzionale del 2001. Non dobbiamo dimenticare come questo Governo e la maggioranza parlamentare abbiano rispettato la norma contenuta nella finanziaria

Riteniamo che il rispetto sostanziale di questa norma debba essere ascritto in positivo all'attuale Governo e a questa maggioranza parlamentare. Salva la necessità di avere un Ministro del turismo per le note ragioni, in carica alla Presidenza del Consiglio, è tornata attuale l'estrema necessità, anche alla luce di quanto sta avvenendo, dello stabilire nuovamente l'autonomia del Ministero della salute, scorporando il medesimo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

è chiaro che nell'affrontare ogni testo normativo l'opposizione utilizza una serie di elementi e di strumenti

fa parte comunque degli strumenti dell'opposizione e della dialettica parlamentare. Le motivazioni argomentate dal collega D'Alia reggono in modo molto labile, al punto che troviamo ripetuto in

uscivamo infatti da una compagine di Governo tanto larga e tanto rigonfiata - parliamo dell'ultimo Governo Prodi - per mantenere equilibri politici estremamente instabili,

Non stiamo parlando di una piccola riduzione, non è stata fatta una rivisitazione, anche in funzione di un risparmio e di una migliore allocazione di risorse: è stato operato un taglio draconiano! Non c'è dubbio però che questo assetto di Governo nel tempo ha manifestato qualche sbavatura; se i numeri sono così bassi e se il Governo è chiamato a rispondere ad una pluralità di stimoli, di domande, di interventi in funzione dei relativi Dicasteri, dovendo Ministri e Sottosegretari

probabilmente ha comportato qualche sfilacciatura, qualche disguido operativo. Avere un Ministero che si occupa direttamente dei problemi delle Regioni significa esattamente il contrario di quanto sollevato nella questione pregiudiziale, perché va nella direzione di migliorare e di non appesantire o addirittura schiacciare le Regioni con nuove attribuzioni attribuzioni a livello centrale. Agevoliamo, viceversa, le Regioni, con un unico interlocutore che non avrà neanche bisogno di interfacciarsi e di passare attraverso il Ministero del *welfare*, realizzando una presa diretta Regione-Stato.

obiezioni. Se guardiamo poi la funzionalità e l'assetto, non possono cambiare, seppur minimamente, rispetto alle funzioni che già svolgeva

noi per primi nel dibattito per la costituzione del nuovo Governo avevamo chiesto con forza l'istituzione del Ministero e, quindi, di non cambiare l'assetto che era stato dato dalla già richiamata legge Prodi

un conto è dire che non è più possibile pensare che il comparto della sanità sia ricompreso all'interno di un megaministero, ma debba avere una sua specificità e autorevolezza,

abbiamo una vera e propria violazione delle competenze regionali in termini di programmazione sanitaria

tutti con curiosità - a questo punto non dico più con speranza - le norme applicative in materia fiscale ed economico-finanziaria.

cosa succederà nella riorganizzazione del Ministero cui vengono sottratte queste competenze.

Collega Ferrara, i Parlamenti non si reggono sulle cose interessanti dette dai parlamentari, ma sul loro diritto di parlare. Quindi, eviti di fare commenti di merito su questo tema, che sono disdicevoli!

il senatore Ferrara ci ha deliziato con le sue riflessioni approfondite. ADAMO *(PD)*. Gli faccia pervenire una camomilla in formato gigante! Come dicevo,

a 63. Le ragioni per cui si pongono dei dubbi sui costi sono anche queste. Non si sta andando a costituire un nuovo Ministero,

«programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali»; sono sostituite dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, Cosa vuol dire? Significa che il Ministero deve intervenire nella discrezionalità tecnica di attuazione degli

ma personalmente non capisco. Il dubbio è che il Ministero voglia entrare nel merito di come le Regioni, nella loro autonomia costituzionale, decidono, fatto salvo il coordinamento nazionale della programmazione sanitaria, e quindi i livelli minimi. In realtà decidono loro. Si può tornare indietro

sono del tutto pleonastici in questo caso. Vogliamo amplificarli? Vogliamo dire che il Ministero dell'economia interviene nella procedura di rientro

la sanità regionalizzata non funziona. Vi assumete la responsabilità di dirlo e coerentemente operate delle scelte. Se così non è, questa partita va modificata, come va modificata l'espressione

avrebbe avuto come conseguenza l'indebolimento dell'azione programmatica e di gestione del rapporto con le Regioni che, non dimentichiamolo, sono quelle oggi deputate ad attuare le politiche sanitarie sul territorio con un'ampia autonomia sia gestionale che, in parte, anche di spesa. I fatti poi ci hanno dato ragione, certo, non solo perché è mancata l'istituzione del Ministero della salute (vi sono state evidentemente delle scelte politiche) ma perché si è rotto il patto con le Regioni e si sono accentuate con le Regioni le conflittualità, tanto che oggi non sappiamo se il nuovo Patto per la salute sarà sottoscritto alla data prevista del 15 ottobre, con un ritardo di un anno, vorrei ricordare. Tutti gli aspetti di politica sanitaria di questo Paese sono apparsi sempre più sfumati: il Libro verde o il Libro bianco dove, oltre al fatto che non ne condividiamo gli orientamenti, preoccupante è il poco spazio che è stato dato a tematiche così importanti come quelle della salute. queste tematiche, alla fine, dove sono finite? In provvedimenti che trattavano materie diverse quindi, sono apparsi scoordinati tra loro, non legati ad obiettivi di salute per il Paese e quindi ad un progetto Questo ha creato anche molto disagio nel mondo della salute nel nostro Paese tra gli operatori, tra chi deve programmare ed attuare quelle politiche. Inoltre, abbiamo di fronte vorrei ricordarlo - una emergenza abbastanza complessa. Il rischio di pandemia dell'influenza A non è ancora scongiurato e questo metterà a prova tutta la struttura sanitaria del Paese, anche se non dovesse trasformarsi in qualcosa di più grave rispetto all'attuale andamento benigno che ha questo tipo di influenza. Quindi, tutto questo dimostra come sia necessaria una forma di coordinamento ed una forte autorevolezza nel rapporto con gli organismi internazionali che si occupano della salute in un mondo globalizzato. Non a caso, tutti i Paesi europei hanno il Ministero competente; anche gli Stati Uniti, dove sappiamo che gran parte dell'intervento sulla salute è privatizzato. Come Come veniva ricordato, abbiamo valutato in modo positivo questo provvedimento anche se alla sua lettura alla sua lettura sono sorti tutti i dubbi che prima venivano ricordati, perché abbiamo visto le molte modifiche rispetto alle competenze precedentemente previste per questo Ministero. Queste modifiche vanno nella direzione di ampliare delle competenze tecnico-programmatiche. Questo non è molto chiaro nel provvedimento. Però, sorge chiaramente il dubbio quando si parla di possibilità del Ministero di intervenire sulle questioni tecniche, perché questo rischia di dare veramente un colpo all'autonomia tecnico-organizzativa, oltre che programmatica, delle Regioni. Il governo del sistema sanitario nazionale è una prova di federalismo per questo Paese, perché è già in essere da tempo l'autonomia delle Regioni, non solo dalla modifica del Titolo V, ma ancora prima, dal decreto n. 502 del 1992 e successivi, che hanno dato alle Regioni una forte possibilità organizzativa e di intervento. Successivamente, nella sperimentazione, le Regioni sono diventate ancora

non solo per le singole Regioni, è un compito gravoso ed importante che spetta al Governo nazionale, e quindi ad un Ministero, coordinare. Non è certo questione di spesa sanitaria; vorrei ribadire che non si può limitare l'intervento nel campo della salute sempre adducendo la spesa sanitaria. Se è vero che la Corte dei conti

limitare l'intervento e la qualità del nostro sistema. Si tratta invece di essere molto esigenti nel chiedere il rientro rispetto alle situazioni di deficit che si sono determinate e soprattutto di perseguire un'azione che non sia solo quella di un taglio della spesa o di riversare sui cittadini il costo di questi deficit*,* prevedendo ulteriori addizionali IRPEF o istituendo dei *ticket*. Vanno attuate politiche per riorganizzare e riqualificare i servizi, affinché l'uscita dalla crisi che stanno vivendo queste Regioni porti anche ad elevare i diritti dei cittadini e la qualità di quei sistemi sanitari

e non sia anche un fattore di benessere e di salute che incide sull'economia del Paese. Questo credo sia inaccettabile, non solo perché l'Europa ci dice che salute e benessere sono la ricchezza di un Paese e una ricchezza per l'Europa, ma anche perché, vorrei ricordarlo, importanti economisti ormai sostengono che il prodotto interno lordo non può essere basato solo su fattori economici ma deve riguardare anche fattori di benessere, di salute e di vivibilità delle nostre città.

continuamente al coordinamento del Ministero del tesoro. Esiste una sede collegiale dove i Ministri si ritrovano ed è il Governo; in quella sede si discutono le compatibilità, ma alla base di strategie più generali di qualità del nostro sistema economico e sociale e di convivenza civile. Se si vuole realizzare delle economie le si facciano, ad esempio, riducendo il numero dei Sottosegretari. Oltretutto, questo provvedimento è diventato anche una scorciatoia per allargare il numero dei Sottosegretari di altri Ministeri;

poste anche nell'intervento che mi ha preceduto, non solo riguardo al numero dei Sottosegretari ma anche all'allentamento del blocco delle assunzioni del personale dirigente e non,

della salute così come per un no. Fino ad oggi nel Governo Berlusconi avevano prevalso le ragioni del no ed infatti, a tutt'oggi, siamo senza un Ministro ma con un Vice Ministro della salute. Le buone ragioni per il no possiamo riassumerle in una battuta. L'evoluzione del modello di organizzazione sanitaria in Italia negli ultimi trent'anni mostra una tendenza al decentramento e al federalismo sanitario che, quindi, vede come naturale conseguenza

la necessità di avere un Ministero - evidentemente prevalgono, anche nella maggioranza, le buone ragioni per avere un Ministro della salute.

prevedendo comunque all'interno un Dipartimento di salute con un responsabile senza rango di Ministro, ma di Vice Ministro o di Sottosegretario. Comunque, anche in questi Paesi la situazione si è sempre alternata. Pensiamo poi che siamo in Italia, dove abbiamo un sistema sanitario nazionale, in cui la salute è uno dei maggiori obiettivi - così come in ogni Paese - e la sanità è uno dei settori più importanti: vale da noi il 9 per

dei cittadini. Di più possiamo dire che non soltanto la salute è un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione, ma è un diritto umano e che quindi in quanto tale va tutelato: queste sono le buone ragioni che ci fanno propendere per avere un Ministro

è l'accorpamento di due disegni di legge. Da una parte, c'è l'istituzione del Ministero della salute e, dall'altra, esso utilizza le buone ragioni per l'istituzione del Ministero della salute per ampliare il numero dei componenti del Governo.

evita, nel caso, di mischiare le due questioni, di chiedere cioè un voto sul Ministero della salute, così importante e, con l'occasione, rifilare un paio di Sottosegretari

sottolineato in più emendamenti dell'opposizione - alcuni li abbiamo presentati anche noi come delegazione radicale - che rilevano l'assoluta

potrebbe apparire pleonastico, dato che il Consiglio dei ministri è organo collegiale e, quindi, tale concerto deve sempre essere previsto quando si prendono delle decisioni. Se le preoccupazioni fossero semplicemente di tipo tecnico-economico, basterebbe specificare e sapere che ogni decisione di tipo economico è, fra l'altro, sempre sotto il controllo e le valutazioni della Ragioneria generale Stato; invece, scriverlo nero su bianco nella legge sembra voler specificare che si va a creare un Ministero della salute che però è sostanzialmente dipendente dal Ministero dell'economia

buone ragioni per istituire un Ministero della salute, è perché esiste un sistema sanitario nazionale. Vi sono certamente le competenze, la forza e il governo delle Regioni, ma il sistema sanitario è nazionale e il diritto alla salute è riconosciuto nella Costituzione. Sicuramente,

la valutazione indipendente di tutti i servizi e delle strutture del sistema sanitario, nonché l'organizzazione dell'informazione sui risultati delle valutazioni in modo facilmente accessibile ai cittadini.

da chi eroga i servizi, vive e ha interessi nella sanità, perché vediamo bene quanti, di che tipo e di che portata siano gli interessi della sanità e non tanto della salute dei cittadini. Questi strumenti dovrebbero essere forniti ai cittadini in maniera tale che essi possano scegliere le strutture di cura ed i percorsi terapeutici, conoscendone anche la reale efficacia. Insomma, è il solito sistema di valutazione, di informazione di scelta consapevole dei cittadini. È quindi riportato anche in questo ambito il principio più generale e fondativo di qualsiasi società liberale, quello del conoscere

signor Vice Ministro, la costituzione di un autonomo Ministero della salute è un atto intelligente. Parlando con un profilo meno federalista e meno regionalista, io affermo che

né l'organizzazione del servizio sanitario né la ricerca all'interno di un ambito squisitamente regionale o di piccola area. Credo, pertanto, che il profilo di un Ministero che sappia programmare tenendo conto di queste realtà sia una necessità non differibile. Mi sta molto a cuore un sistema sanitario nazionale che oggi ho difficoltà a definire tale; si tratta di un sistema sanitario che è costituito dalla sommatoria dei sistemi delle singole Regioni e i cui esiti sono una media che non sempre brilla. anche di quelli conseguiti dalle Regioni migliori. Credo che l'intervento di un'istituzione, ripeto, autonoma e autorevole possa ridare all'aggettivo nazionale un suo significato più pregnante.

Credo che dovrebbe essere compiuta una fatica, forse nuova, ma - mi pare - anche abbastanza interessante dal punto di vista politico. Tutti gli studi ci dicono che i determinanti non medici di salute sono ben più significativi di quelli medici rispetto alla possibilità dello star bene

anni; questo è vero a bocce ferme o se non accadono altre cose. Noi immaginiamo che dovremmo fare di tutto perché questo accada e perché si arrivi a quell'età stando meglio che si può. Sappiamo benissimo però che l'ultimo tratto sarà difficile se non saranno intervenuti quei determinanti non medici (l'educazione, l'istruzione,

questo sia un problema che dovrebbe in qualche modo anche riguardare il profilo economico, che non vedo in questo momento così significativo. Non vorrei che questo legame non virtuoso determinasse una scarsa autonomia e una scarsa autorevolezza e impedisse fin da subito di raggiungere i risultati più facilmente raggiungibili, ovvero un riequilibrio di servizi nel nostro Paese tra Regioni virtuose e meno che necessitano di una politica forte a livello nazionale, di una programmazione che da subito faccia spendere bene le risorse disponibili. Questi risultati sono ottenibili immediatamente attraverso autorevolezza e autonomia. Sono soprattutto importanti quelli che richiedono una lunga gittata di pensiero e fantasia

Allora, se l'obiezione è che tutto questo riguarda un futuro lontano, se l'obiezione è che sostanzialmente dobbiamo preoccuparci di far tornare i conti subito, perché è più importante di quanto sia pensare alla salute del Paese nei prossimi venti o trent'anni, credo che invertiamo l'ordine dei fattori, perché a noi oggi deve preoccupare proprio questo. Credo che come legislatori dobbiamo immaginare che nel futuro del nostro Paese ci debba essere un futuro di salute, e questo lo si fa se oggi si mettono in atto alcune iniziative. Abbiamo imparato in questi anni, anche noi medici, a far di conto, e oggi ci chiediamo più facilmente - e sappiamo dare anche qualche risposta quanto costiamo, quanto spendiamo. Lo abbiamo fatto con un po' di riluttanza. Ma c'è un costo che non sappiamo calcolare, e che puntualmente la storia ci presenta (si potrebbe già misurare rispetto al passato), ed è quello dell'inazione: non fare costa, non prendere iniziative rispetto ad un futuro che entro certi limiti si conosce costa. Se oggi non mettiamo in atto una politica della salute in grado di prevenire la cronicità

mancanza di rispetto verso il proprio disegno, verso la propria capacità di intuire quel che si deve fare nel settore che si conosce. conosce. Dovrebbe esserci una pari dignità, che oggi non riesco a leggere in queste pagine. Quindi, quell'atto intelligente, che ritengo sia la costituzione del Ministero, va compiuto fino in fondo, con grande autonomia, con grande autorevolezza, con la dignità che viene chiesta a chi assume su di sé la responsabilità di disegnare in termini di salute il futuro del Paese e di quella cittadina che nascerà oggi o domani, con un'attesa di vita che vuole essere anche l'attesa di una buona qualità della vita. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli senatrici e senatori, finalmente! C'è voluto un anno e mezzo e un'emergenza sanitaria come quella che ci stiamo preparando ad affrontare con l'epidemia di influenza A, ma finalmente il Governo si è deciso a riconoscere un grave errore ed a porvi rimedio. Con il Governo Berlusconi nel 2008, per la prima volta nella storia della Repubblica, l'Italia ha cancellato il Ministero della salute e con esso un coordinamento centrale e una figura di riferimento autorevole per i problemi dei pazienti, dei medici, degli infermieri e di tutto il mondo della sanità. È vero che da alcuni anni molte competenze sono state trasferite alle Regioni, ma è altrettanto vero che un coordinamento nazionale è sempre stato considerato essenziale per salvaguardare i princìpi di omogeneità su tutto il territorio nazionale e di equità

significa che si riconosce ad un determinato settore un'importanza strategica, cruciale per la vita dei cittadini e per il buon funzionamento dello Stato. E io penso, come mi avete più volte sentito ripetere, che la salute delle persone sia un fatto strategico importantissimo per chi ha la responsabilità di governare un Paese.

Facendo i miei migliori auguri di buon lavoro a chi sarà scelto per guidare il Dicastero della salute, auspico che d'ora in poi il nuovo Ministro si batterà per un più adeguato finanziamento del settore della sanità pubblica e non accetterà i tagli indiscriminati e disastrosi decisi da altri Ministri. Penso ad esempio ai fondi necessari per la modernizzazione della rete ospedaliera: in Italia abbiamo poco più di mille ospedali, 600 dei quali costruiti prima del 1940. Serve un finanziamento di dimensioni epocali e sappiamo tutti che è davvero necessario. Mi aspetto inoltre che l'Italia possa iniziare a giocare un ruolo autorevole e riconosciuto a livello internazionale dagli altri Ministri della salute europei ed extraeuropei nel compito della prevenzione di malattie che pongono problemi planetari: basti pensare all'influenza o al bioterrorismo. I compiti che aspettano il nuovo Ministro sono davvero ardui, delle vere emergenze, che vanno dalla sicurezza degli ospedali al controllo e alla valutazione delle prestazioni e dei professionisti nel pubblico e nel privato, alla gestione del divario enorme tra la sanità del Nord e quella del Meridione, che arretra sempre di più e nei fatti priva i cittadini del Sud del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione. Mi permetto di dare un suggerimento a chi assumerà l'incarico di Ministro: provi a fare un viaggio in aereo a Lamezia Terme e a guardare, appena uscito dall'aeroporto, l'enorme tabellone dove è scritto: «Voli sanitari privati per pazienti».

che è essenziale nella sanità moderna: quella di introdurre nel sistema sanitario la cultura della valutazione. Servono strumenti per valutare: serve un organismo snello - uno solo - con ampi poteri di intervento, che valuti periodicamente l'operato di *manager* e dirigenti sanitari, come avviene in molti altri Paesi. Per rendere efficiente il nostro sistema sanitario vanno controllati e valutati la qualità dei servizi, la sicurezza, gli sprechi dal punto di vista clinico ma anche gestionale, e, seguendo criteri identici, dovrebbero essere valutati sia il servizio pubblico sia le strutture private. C'è un grande lavoro da compiere, e per questo esprimo la mia soddisfazione per l'istituzione del Ministero della salute.

Resterei sorpreso se davvero il Partito Democratico - per disavventura, devo dire - dovesse scegliere alla propria guida un siffatto segretario, che ha dichiarato che per la prima volta un Governo della Repubblica, il Governo Berlusconi, ha cancellato il Ministero della salute. Neppure sa che il provvedimento è stato assunto dal Governo Prodi con un decreto-legge *(Applausi dal Gruppo PdL)* e che il Governo Berlusconi ha dovuto necessariamente, trattandosi di un decreto-legge, a meno di non poter nominare Ministri, regolarsi come ha fatto. C'è di più. neppure sa che l'abolizione di questo Ministero è nella tradizione della sinistra di governo italiana, che l'aveva già abolito in conseguenza dei provvedimenti di riorganizzazione Bassanini e che il Governo Berlusconi una prima volta lo aveva reintrodotto con un provvedimento, tanto che il primo Ministro della salute della Repubblica italiana - buon per lui! - è stato il buon Francesco Storace. C'è, in sostanza, una mancata conoscenza conoscenza della realtà italiana e un capovolgimento nell'addebito di responsabilità davvero sorprendente, che dimostrano indirettamente in quali condizioni versa oggi il Partito Democratico nella sua ricerca di *leadership*.

Esso nasce come risposta alla scellerata decisione del centrosinistra che, senatore Marino, non è casuale, ma di origine culturale. Essa risale non soltanto alle decisioni di Bassanini,

riguardante l'inserimento del concetto di sanità all'interno del diritto alla salute come diritto che appartiene a tutti gli italiani. Tanto per rinfrescare la mia memoria e quella del senatore Marino, Marino, dico che il delitto più grande commesso dal centrosinistra non è stato quello di attribuire in maniera scoordinata e senza un punto di riferimento di carattere generale la sanità alle Regioni perché in questo potremmo dire che non c'era nulla di grave, tant'è che nella riforma che è stata poi bocciata, purtroppo, dagli italiani

assegnata alle Regioni la competenza anche in materia di salute, facendo diventare un diritto costituzionalmente garantito materia di legislazione concorrente,

e giustamente richiamata dal senatore D'Alia, ma non perché la condivida. Conosco infatti benissimo il pensiero del collega D'Alia, peraltro intervenuto nella cosiddetta riforma di Lorenzago per eliminare questa degenerazione, questa stortura, questo delitto posto in essere dal centrosinistra,

salute, senatore Marino, appartiene alla sua storia, ad una storia che fa concludere il riferimento unitario su questo tema. Ma la salute, come lei ben sa perché l'ha espresso tante volte, non può essere spezzettata. La salute appartiene a tutti, e vi è di più: è ancora più grave che in questa proposta di riforma soltanto *ex post* si stabilisce la possibilità della Corte costituzionale di intervenire nel caso in cui vi sia una violazione dei livelli minimi essenziali. Si sono talmente sforzati di recuperare un minimo di coordinamento unitario, dopo il delitto commesso, da chiamare in causa i livelli minimi essenziali rispetto a un diritto che, invece, è tipico e costituzionalmente garantito nell'articolo 32 della Costituzione. In conclusione, a me non interessa il dettaglio.

né di dire, come il senatore Gustavino, «è una proposta intelligente, ma..»: è una proposta intelligente, è una proposta valida, perché fa vedere che in questa Italia ancora esistono lo Stato e l'unità nazionale, e che su questo tema occorre un Ministero che esprima punti di vista e decisioni e dia istruzioni e orientamenti, che garantiscano la tutela della salute e ai quali le Regioni si devono adeguare, perché la salute non appartiene alla Regione, ma appartiene al popolo italiano e la tutela della salute appartiene a tutti.

Signor Presidente, spero che la Corte costituzionale avrà modo di esprimersi appieno sull'interpretazione dell'articolo 32 da poco evocata dal senatore Nania, perché mi pare che ne sia stata data una interpretazione non so se dire restrittiva ma sicuramente manipolativa durante il dibattito relativo al testamento biologico,

vuole andare nella direzione già adottata in altri ambiti tanto dalla Camera, quanto dal Senato e fatta propria dal Governo, in particolare dal ministro Brunetta, relativa *in primis* alla trasparenza dei dati che attengono all'amministrazione pubblica e, in seconda battuta, alla possibilità di far valutare al cittadino l'operato dei dipendenti dello Stato e quindi,

L'ordine del giorno di carattere generale che abbiamo voluto presentare va in questa direzione e credo non vi sia modo migliore di illustrarlo che leggerlo: premesso che: la popolazione italiana presenta ottimi valori di salute (fra i migliori del mondo) e partecipa di un buon livello complessivo di sanità, comparabile con quella degli altri paesi di pari sviluppo economico; economico; nel quadro del sistema sanitario nazionale, è però innegabile la presenza di problemi evidenti e misurabili laddove si guardi alla forte disomogeneità dei servizi sul territorio, o a un rapporto mediocre con gli utenti,

ed è in linea con la media dei principali paesi industrializzati. Un ulteriore aumento della spesa sarebbe anzi deleterio perché andrebbe a consolidare le inefficienze e ritarderebbe le soluzioni; soluzioni; in alcuni Paesi (soprattutto quelli anglosassoni), il ruolo del cittadino è visto sempre più come attivo e incidente sul governo del sistema. La vera proposta riformatrice per l'Italia in campo sanitario sarebbe l'introduzione di un sistema di Valutazione-Informazione-Scelta a tutti i livelli del sistema sanitario, trasformando il cittadino-paziente in soggetto attivo e strumento esso stesso di governo del sistema; in questa logica e con questo obiettivo, sarebbe opportuno creare sistemi di valutazione quantitativa indipendente per tutti i servizi sanitari, a tutti i livelli del sistema, rendendo pubblica, semplice e facilmente accessibile l'informazione sui risultati delle valutazioni; tra le proposte operative immediate ed attuabili a breve sarebbe necessario: 1) rendere pubblici curricula, obiettivi, risultati e valutazioni dei Direttori Generali di AO e ASL attraverso la creazione di una anagrafe pubblica digitale; creare un sito web ove i pazienti dei Medici di Medicina Generale possano esprimere il grado di soddisfazione sul proprio MMG, relativamente a puntualità, reperibilità, disponibilità al dialogo, completezza delle informazioni, organizzazione;

rendere possibili comparazioni e risultati delle valutazioni sia via internet che fisicamente in loco; 4) definire un vero sistema di valutazione indipendente della reale efficacia delle cure e dei farmaci

ed un sistema di informazione sui risultati che sia facilmente accessibile a tutti i cittadini». Ripeto che tutto ciò è in linea con quanto si sta iniziando a fare per rendere non soltanto più trasparente - cosa che già di per sé rappresenta una nota di merito - l'amministrazione pubblica, ma anche per far conoscere

è poi l'esigenza di sottolineare con forza - mi auguro che chiunque sarà chiamato a svolgere le funzioni di Ministro lo faccia - i temi della sicurezza alimentare. Abbiamo combattuto per anni con il presidente Berlusconi, nel Governo 2001-2006, per creare a livello nazionale un'Agenzia per la sicurezza alimentare,

cui sento parlare poco. La Commissione ha ricevuto la relazione annuale al Parlamento, ma mi sembra di capire che su questa vicenda vi sia bisogno di un rafforzamento dei poteri ed anche di una modifica della Commissione a livello centrale che riveda nel Dicastero della salute e nel Ministro organi di riferimento importanti.

L'aver affidato, con la modifica al Titolo V, che passò per quattro voti, alle Regioni la gestione e l'organizzazione della sanità non è più sufficiente.

qualcosa che non funziona. Ecco, dunque, la funzione importante che può svolgere il Ministero della salute, che ha richiamato spesso e volentieri e si è dovuto attaccare ai LEA per fare in modo che le Regioni ragionassero in maniera diversa.

qualunque Ministro della salute che voglia definire fino in fondo un percorso importante sui temi della ricerca e destinare ad essa fondi adeguati. Solo con la ricerca si entra in Europa e nel mondo; solo con la ricerca si diventa un paese di serie A e non si scade a livelli di retroguardia.

Siamo andati a verificare come una politica del farmaco sostenuta a livello nazionale, in un'intelligente raccordo con la Regione, nel caso specifico la Toscana, abbia dato risultati importanti. a livello nazionale ed europeo, che un'azienda potrà assumere con l'indotto anche 1.000 persone e rilanciare un sistema che faccia di quell'azienda farmaceutica il punto di riferimento per la produzione di insulina a livello europeo è un fatto politicamente rilevante ed importante, Anche con riferimento alla politica del farmaco vorrei ricordare a me stesso e ai colleghi quanto è stato fatto nel 2003-2004 con l'accordo di programma,

Questa è la strada che dobbiamo imboccare se vogliamo che l'Italia, come oggi, sia il terzo Paese a livello europeo che consuma e produce farmaci.

far capire ai cittadini che stiamo lavorando per la loro salute e che l'articolo 32 della nostra Carta costituzionale non è una norma qualsiasi, ma è quella che garantisce la tutela della salute di tutti i cittadini.

Bassanini 1 aveva previsto l'unificazione di quei Ministeri. Voglio ricordare a me stesso, ma anche ai colleghi, la necessità sentita da tutti coloro i quali

precisa perché il Presidente era troppo impegnato nella sua personale campagna elettorale. Questo però non è il problema dell'istituzione del Ministero.

l'amico Ferruccio Fazio da Sottosegretario è diventato poi Vice Ministro, proprio per dargli la possibilità di sedere in modo paritario con i Ministri della salute europei. Voglio ricordare a me stesso

a livello nazionale ed internazionale. Penso ai LEA e a tutto ciò che nel campo dei LEA un Ministero della salute deve rivedere con intelligenza, comprendendo quali sono oggi le istanze e le richieste dei cittadini che hanno bisogno di interventi concreti sul piano della salute. Non quindi una contrapposizione dovrà avere questo Ministero nei riguardi delle competenze specifiche delle Regioni che nominano i direttori generali delle singole aziende, ma una collaborazione attiva che permetta di conoscere realmente il ruolo che questi direttori generali andranno a svolgere, le rispettive competenze e ciò che dovranno fare, fare bene, proprio in funzione della scelta per la sanità. Lo scorso lunedì, partecipando ad un dibattito promosso da realtà sanitarie qui al Senato, il collega Gustavino nel suo intervento ribadiva la necessità di arrivare oggi ad un consenso il più largo possibile affinché questo Ministero abbia poi le spalle coperte da un preciso impegno parlamentare,

che ha bisogno, secondo noi, proprio di questa attività di coordinamento. E a chi in questi giorni e prima di questo dibattito ha evidenziato che siamo

occhio di riguardo e manifesta la volontà politica di non cancellare un ruolo di coordinamento che il Ministero della salute deve tornare ad avere, anche per non contrapporre Regione a Regione sul sistema di assistenza sanitaria.

che abbia a cuore l'interesse della salute pubblica.

Credo che, anziché aprire dibattiti, come spesso è accaduto in questa e in altre legislature, sui drammi della sanità nazionale e la gestione di alcune Regioni che hanno provocato buchi di bilancio e sperpero di risorse (rispetto ai quali si è dovuto provvedere,

ma che non si neghi a un'apertura nel momento in cui il Parlamento ritenesse di cambiare - come pure aveva fatto tra il 2001 e il 2006 - l'articolo 117 della Costituzione, se ciò avverrà in questa legislatura. In molti avevamo pensato che fosse la legislatura giusta; molte circostanze del dibattito politico ci fanno però capire che in questo momento il clima esterno difficilmente si presta a larghe intese per cambiare la Costituzione, e io sono fra quelli convinti che la Costituzione non si cambia a colpi di maggioranza. Siamo comunque pronti a prendere atto che quando le Regioni avranno maggiori poteri e anche maggiori responsabilità, a cominciare dall'attuazione del federalismo fiscale, si potrà addivenire ad una normativa diversa, che tenga conto del cambiamento del rapporto istituzionale tra le Regioni e lo Stato centrale, quando questo sarà sancito dalla Costituzione. Ad oggi ci sembra meglio operare preventivamente, con un controllo accurato, e non dopo che il guaio da molte parti è stato fatto. Lo dico io che provengo da una Regione meridionale che spesso questo guaio ha finito per procurarlo e che sta cercando faticosamente di rimettersi in cammino nella giusta direzione. La seconda osservazione che è stata fatta concerne l'aumento dei Sottosegretari, ai quali già qualcuno, nel parlare, attribuisce le deleghe. Noi stiamo approvando una legge in cui si dice che il numero dei membri del Governo può raggiungere le 63 unità. Non stiamo fissando per legge quale sarà la delega dei nuovi Sottosegretari; toccherà al Governo, un atto proprio, disciplinare la sua organizzazione, ma sfido chiunque in quest'Aula, sulla scorta dell'esperienza fatta in questa legislatura nelle Commissioni, a dire che non si è dovuto interrompere o far slittare di un giorno una seduta,

ognuna per conto proprio le leggi, a cominciare dalle Conferenze dei Capigruppo, che quando si riuniscono hanno bisogno della presenza di un rappresentante del Governo (e in questo caso il Ministro per i rapporti con il Parlamento non ha nessuno che possa

Dire questo significa evidentemente non volere che il Parlamento funzioni correttamente. La terza osservazione la voglio fare, senza polemica, rivolgendomi al professor Marino,

Ma la cancellazione del Ministero della salute nasce dal cosiddetto Bassanini 1, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che fissa in 12 il numero dei Ministeri e istituisce il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

riprendendo i contenuti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Questo Governo, dopo aver dovuto attuare il dispositivo della finanziaria, si è reso conto esattamente

ad un tentativo sbagliato che era stato fatto in questo Paese. Tengo a dire che questo tentativo sbagliato non l'aveva fatto la parte politica a cui appartengo; tengo a dirlo perché abbiamo avuto da sempre questa visione e averla oggi tutti insieme è un fatto positivo che registro con favore. Per il resto, credo che il dibattito sia stato ampio, sereno e articolato; esso ha consentito di misurarci con una serie di convergenze e alcune divergenze contenute negli emendamenti. Considero comunque un fatto positivo

per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la pianta organica cui fa riferimento il comma 8 sia quella di fatto di fatto al 30 settembre 2008, secondo quanto stabilito dall'articolo 74, comma 5, del decreto-legge n. e nel presupposto che dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non debba derivare alcuna revisione dei trattamenti economici in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti. Rileva altresì la necessità di acquisire più puntuali elementi informativi circa la concreta realizzazione dei risparmi di cui al comma 9, nel presupposto che essi siano finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 247 del 2007. Riguardo alla previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, punto osserva che l'intervento dello Stato, relativo ai piani di rientro regionali, deve essere inteso non soltanto in termini di intervento di carattere finanziario, ma piuttosto in attività di coordinamento, controllo e supporto nella redazione dei piani medesimi».

parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.101, 1.105, 1.106, 1.103, 1.108 e 1.0.1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

per quanto riguarda il primo problema, sarebbe giusto parlare di due sistemi sanitari (quello delle regioni del Nord-Centro e quello delle regioni del Sud-Centro), per il secondo tutti gli indicatori (anche l'Euro Health Consumer Index) mostrano che riguarda l'intero sistema nazionale; 3) creare sistemi di valutazione di strutture e servizi, per renderne pubblici i risultati e quindi la richiesta di applicazione del sistema di valutazione del NHS (con eventuali modifiche e integrazioni) a tutte le strutture del sistema sanitario italiano; rendere possibili a definire e realizzare, in accordo con le Regioni, un sistema di valutazione indipendente delle diverse tipologie di servizi sanitari erogati ai cittadini nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed un sistema di informazione sui risultati che sia facilmente accessibile a tutti i cittadini.

Come avevo già spiegato nel mio precedente intervento, tali emendamenti tendono sostanzialmente a intervenire su tre questioni. Il primo

Ministro. È ovvio che un Ministro non può essere onnipresente: vogliamo dunque concedere un Sottosegretario? Arriviamo a 61. Gli altri due Sottosegretari a che cosa servono? Non servono al Ministero della salute perché, come abbiamo visto in precedenza, il provvedimento separa completamente il numero dei componenti del Governo dall'assetto del Ministero. Servono ad altre necessità della Presidenza del Consiglio.

Non vogliamo sollevare una questione di tipo demagogico, sostenendo che aumentando il numero dei Sottosegretari si aumenta inutilmente la spesa, ma abbiamo il diritto di sapere cosa vuol fare il Presidente del Consiglio di due nuovi Sottosegretari.

estese ed esorbitanti rispetto alle competenze regionali ma, nello stesso tempo, limitate e sottoposte al concerto

Per gli equilibri politici creiamo un Ministro che, però, non avrà le funzioni di indirizzo e coordinamento della politica sanitaria, ma solo di controllo della spesa attraverso il concerto

Come diceva giustamente la collega Bassoli, noi riteniamo che in questo modo non stiamo rispondendo pienamente all'esigenza che poneva anche il senatore Marino, quando con forza ribadiva le ragioni della nostra richiesta del Ministero della sanità, ma stiamo istituendo un Ministero

dalla sorveglianza speciale (che gli viene apposta con l'espressione «di concerto» per ogni decisione) del Ministero dell'economia sarebbe un buon risultato

sia votato da tutti i senatori di quest'Aula perché questa sarebbe proprio la volontà del Senato.

anche perché il Ministro per i rapporti con il Parlamento possa avere un Sottosegretario, ci mancherebbe altro, questo va nell'organizzazione delle cose. Per me il numero dei componenti potrebbe anche essere allargato a 83;

di posti di livello dirigenziale generale e non, nonché procedere all'assunzione di personale non dirigenziale, sia pure nei limiti delle norme vigenti in materia. A

Propone che sia competenza del neonato Ministero anche il «monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sulla quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento». fare una riflessione a sostegno di tale emendamento. Noi abbiamo una totale incapacità di riformare gli assetti costituzionali. Il collega Nania nel suo intervento stamattina ricordava un voto di maggioranza per la riforma del Titolo V della Costituzione, una maggioranza di pochissimi numeri che in realtà trasformava - appunto a colpi di maggioranza - un'intesa raggiunta all'unanimità nelle Commissioni precedenti (due errori uno dopo l'altro), e una riforma costituzionale, ancora a maggioranza, che poi è stata smentita dal *referendum* (altri due errori uno dopo l'altro). Mi chiedo quindi se, quando si parla di regole, di assetti costituzionali, di federalismo fiscale, di equilibrio tra Regioni e Stato, di competenze di un Ministero, non valga la pena sommessamente di tentare di trovare un'intesa nel Parlamento che coinvolga maggioranza e opposizione. In questo caso segnalo ai colleghi che è in atto una curiosa trasformazione costituzionale, che non ha però alcun riferimento e alcun confronto giuridico. Mezza Italia è commissariata in sanità:

Abbiamo due Italie, non c'è nessuna norma costituzionale che lo dice: un'Italia in cui la sanità è direttamente e strettamente competenza delle Regioni, senza coordinamenti e indirizzi nazionali, e un'Italia in cui ci sono i commissari del Governo. alle questioni economiche e di bilancio sulle quali avvengono i commissariamenti, il disegno di legge al nostro esame è molto povero: si dice che il Ministero che nasce dovrà concertare tutto con il Ministero dell'economia. Si discuterà in un altro momento con il Ministro dell'economia di quali politiche servono per la sanità. 1.13 (testo 2) segnala l'esigenza che forse non è solo sulla compatibilità dei bilanci che occorre una funzione dello Stato in materia di tutela della salute della popolazione: c'è un dritto dei cittadini italiani a vedere garantiti i propri livelli di sicurezza individuali, di salute, di prestazioni sanitarie. Dunque, l'emendamento propone che sia il Governo a svolgere il monitoraggio dei livelli di assistenza, Regione per Regione. Vogliamo esprimerci brutalmente? Ci sono tassi di mortalità maggiori da Regione a Regione per la cattiva assistenza erogata. Perché non è compito del Governo e del Parlamento ragionare, discutere, intervenire? Il rapporto con le Regioni non può che essere solidale di fronte al fatto che ci prendiamo carico del diritto alla salute di tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalle Regioni in cui essi risiedono. Dunque, perché non fare quello che fa uno Stato federale come gli Stati Uniti d'America, cioè la valutazione della qualità assistenziale con la garanzia dei livelli di assistenza per ogni cittadino? Perché non farlo, visto che lo si fa in Inghilterra? L'emendamento propone questo: una funzione dello Stato - in uno Stato organizzato in cui non si discutono le competenze regionali in termini di programmazione e gestione dei servizi - che non è soltanto quella di tenere a bada i conti, ma anche quella di curarsi del diritto alla salute

una norma avulsa in un provvedimento che si occupa di altro. Ho spiegato nel corso della replica quali sono le ragioni complessive di questo piccolo aumento. Non tocca a me, né a noi essere attribuiti i Sottosegretari: questo fa parte dell'organizzazione di lavoro che si dà il Governo, di cui risponde al Parlamento quando si presenta con la sua compagine per chiedere la fiducia.

Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, la questione del Ministero della salute offre un quadro davvero problematico, in cui non è semplice distinguere i pro e i contro. Analizzerò alcuni elementi non univoci che possono costituire motivi di incertezza. L'obiezione alla creazione di un nuovo Ministero può essere fondata sul richiamo alla coerenza semplificatrice e può avere un fondamento. Si può dire alla maggioranza: avevate scelto la via della semplificazione e avevate ridotto i Ministeri e poi, in realtà, una volta iniziata la legislatura avete cominciato a istituirne altri.

tutte le situazioni complesse che si vengono a creare su questo terreno e che, come tutti sanno, hanno una rilevanza finanziaria molto Si può anche dire che le nuove strutture non sono nuovi Ministeri; si può obiettare che la polemica sui nuovi Ministeri mostra una tela smagliata, perché i Ministeri sono senza portafoglio.

di stampa hanno illustrato con dovizia di particolari come la nuova struttura per il turismo debba essenzialmente la propria nascita alla necessità di dare una collocazione all'onorevole Brambilla. Ma il Ministero della salute, che ha invece un portafoglio a suo modo cospicuo, pone altri problemi e ne evoco uno, di bibliografia mentale: per associazione di idee i cittadini quando pensano al Ministero della salute rievocano il pouf di Poggiolini, un direttore generale che nascondeva i proventi dei propri guadagni illeciti nei canapè di casa. Obiezione volgare, triviale? Può essere, però la sanità in Italia si è nutrita di terribili scandali su affari fatti con gli emoderivati falsi, con appropriazioni indebite e falsificazioni. Non è facile distaccare la mente da questa dimensione scandalistica quando si pensa al Ministero della salute. Vi è poi una questione seria ed è la questione istituzionale, che va pesata, perché in quest'atmosfera di nuovo regionalismo intenso, di attribuzione di poteri sostanziali alle Regioni tutti sappiamo che alle Regioni è attribuita la potestà sostanziale sulla spesa sanitaria - l'istituzione di un Ministero della salute può apparire come un potenzialmente va ad incidere sulle autonomie regionali nella loro purezza. Ma, a loro volta, queste autonomie regionali sono tutt'altro che pure e quando si riflette su di esse, senza neanche troppa fatica, è facilissimo andare a trovare enormi deficit che le autonomie regionali hanno creato, in parte grazie alla loro stessa autonomia e irresponsabilità, in parte grazie alle necessità dei casi e e della socialità. Come si fa a colmare il deficit delle Regioni, se i Presidenti delle Regioni vengono nominati commissari speciali per il controllo dei deficit della sanità che le Regioni stesse hanno prodotto? riguardo poteva esserci un barlume di motivazione per giustificare il nuovo Ministero della salute; volendo, si poteva affermare che il nuovo Ministero della salute avrebbe avuto la funzione fondamentale di impegnarsi a coordinare insieme alle Regioni una progressiva riduzione ed un futuro controllo serio del deficit. però questo obiettivo è stato ritenuto troppo ottimistico ed irraggiungibile per poterlo proclamare e, quindi, nelle carte del provvedimento che siamo chiamati a votare non si riesce a trovare un barlume di indicazione che vada L'elemento fondamentale che salta agli occhi è che il Governo e la maggioranza non hanno fornito uno straccio di motivazione per l'istituzione della nuova struttura.

una contrarietà che non deriva dall'esigenza di reintrodurre, non un Ministero, ma le competenze in capo allo Stato sulla tutela del diritto fondamentale alla salute.

dettata dai commissariamenti di numerose Regioni perché inosservanti rispetto ai piani di rientro e, dall'altro, la necessità di coordinare una serie di interventi

un piccolo Ministero, cioè di creare una struttura burocratica che non ha alcuna competenza, perché la Costituzione

Onorevoli colleghi della maggioranza, l'idea di proporre il Ministero della salute testimonia il fallimento di alcuni postulati

non è così: si è verificato nella quotidiana pratica, dal 2001 ad oggi, cioè da quando la Costituzione ha cambiato il sistema delle competenze nel settore della sanità,

e come le scelte importanti riguardanti la salute dei cittadini nei vari territori regionali siano sempre più condizionate da chi ha interessi in questo settore nei diversi territori. ciò è cosa ben diversa dall'esigenza di definire una politica generale in un settore fondamentale che tante risorse economiche assorbe e che tanto grava sulle tasche dei cittadini, sia direttamente che indirettamente, attraverso il pagamento delle tasse. Allora, l'idea di reintrodurre

È un modo che non serve! Bisogna fare qualcosa di più e di diverso. Occorre ricostruire nuovamente il sistema delle competenze statali, attribuendo alle Regioni e alle autonomie locali ciò che realmente possono fare (e non tutto) e riattribuendo allo Stato e al Governo centrale le competenze funzionali competenze funzionali ad un governo nazionale dei problemi della sanità, non solo da un punto di vista squisitamente economico

di tendenziale riorganizzazione e razionalizzazione dei Ministeri, delle funzioni amministrative statali e della spesa pubblica statale, presenta anche un'altra problematicità. È evidente che gran parte dell'esercizio delle competenze del Servizio sanitario nazionale oggi, proprio nel momento in cui tocchiamo con mano quanto costi questo servizio e quanto le Regioni abbiano ampliato la spesa sanitaria non riuscendo più a tenerla sotto controllo,

come rendere più efficace, in questo delicato settore, gli interventi dello Stato e del Governo in favore dei cittadini. Per questa ragione votiamo contro il provvedimento,

di cui all'articolo 117 della Costituzione, oggi, in quest'Aula, trovereste il nostro sostegno e il nostro voto favorevole. Non possiamo però votare un provvedimento che serve solo a creare l'ennesima sovrastruttura (e poi, per chi in qualche modo è superstizioso, il numero 13 non porta neanche tanto bene).

non è certamente un mistero che l'intera azione politica della Lega Nord sia da sempre finalizzata alla modifica dell'ordinamento dello Stato in senso federale e alla devoluzione delle competenze a livello regionale e periferico. In questo caso, però, esprimiamo un voto assolutamente favorevole ad una direzione contraria a questo tipo di impostazione politica, ovverosia al riattivare un Ministero, un qualcosa che va a riaccentrare una competenza già già devoluta alle Regioni. Si tratta di una scelta assolutamente obbligata dai fatti in quanto, pur essendo ormai passati otto anni dalla devoluzione delle competenze in materia sanitaria alle Regioni, dobbiamo registrare che, purtroppo, all'interno del Paese si sono venuti a creare, non un insieme di sistemi sanitari regionali diversificati a seconda delle realtà territoriali, come avrebbe dovuto essere nell'auspicio dello spirito di devoluzione della materia, materia, ma sistemi sanitari regionali che portano ad una prestazione sanitaria troppo diversificata sul territorio nazionale e fondamentalmente con tre velocità diverse. registrano una serie di Regioni, purtroppo ancora troppo poche, che erogano prestazioni sanitarie di assoluto rilievo e di elevatissimo livello non solo in campo nazionale ma in qualche caso con delle eccellenze al livello europeo o addirittura mondiale. Questa è la prima velocità, e l'auspicio è che tutte le Regioni in un futuro possano raggiungere questo tipo di livello. Tuttavia dobbiamo prendere atto che esiste un gran numero di Regioni con una velocità completamente diversa, tanto da non riuscire ad erogare prestazioni. Al riguardo apprezzo tantissimo l'intervento del collega Marino riferito al cartello vicino all'aeroporto di Lamezia Terme. Quello è davvero indice del fatto che in determinate parti del nostro Paese la sanità non funziona e vengono continuamente alimentati ancora questi viaggi della speranza in materia sanitaria da alcune Regioni ad altre. vi è tutto il cosmo rappresentato dalla maggioranza delle Regioni, che si stanno organizzando per avere un sistema più efficiente. Alcune di queste addirittura, anche molto faticosamente e coraggiosamente, stanno

assolutamente indispensabile avere un organismo centrale forte a livello nazionale che possa riuscire a coordinare davvero le Regioni e dare una mano alle parti più deboli a riportarsi in carreggiata in maniera tale che si possa davvero in un futuro - auspichiamo il più breve possibile - riuscire ad avere le stesse prestazioni «dalle Alpi alle Piramidi». Un'altra fondamentale motivazione per cui ritengo indispensabile, o comunque veramente auspicabile l'istituzione di questo Ministero è che alcune tematiche, come è stato ricordato, non riguardano l'organizzazione della sanità ma semplicemente il mantenimento del benessere e della salute. Anche stamattina ne parlavamo in Commissione in sede di audizione del Vice Ministro. Quando abbiamo di fronte le emergenze sanitarie come la pandemia del virus A/H1N1 bisogna avere un coordinamento forte centrale che, da un lato, riesca a sdrammatizzare i falsi pericoli e, dall'altro, possa coordinare su tutto il territorio nazionale degli interventi specifici mirati ed efficaci bypassando le eventuali inefficienze di alcuni sistemi sanitari regionali che purtroppo ancora esistono. Credo che non vi sia veramente molto altro da aggiungere. Ribadisco il voto convintamente e favorevole del Gruppo della Lega Nord all'istituzione del Ministero della salute. avremmo volentieri votato a favore di questo provvedimento, perché penso che la scelta di avere nel nostro Paese un Ministero della salute, come d'altro canto esiste in quasi tutti i Paesi del mondo a garanzia degli standard di salute della popolazione, sia giusta. Tuttavia, il provvedimento che voi ci sottoponete non consente un voto favorevole perché quello che create è un mezzo Ministero ed è una scelta contraddittoria che non è stata sciolta all'interno della maggioranza. E dunque le ragioni di un voto che non può essere favorevole sono semplicissime. In primo luogo, approfittate della giusta esigenza di creare il Ministero della salute per moltiplicare il numero di Ministri e Sottosegretari. Avete criticato molto, e con qualche ragione, il Governo Prodi per un numero troppo ampio di Ministri e Sottosegretari. Ma ci risiamo! La politica ricomincia ad aumentare il numero dei Ministri e Sottosegretari. Umilmente e sommessamente do un consiglio: se si tratta di creare il Ministero della salute ma non si vuole aumentare il numero dei Ministeri, nulla impedisce di abolire l'inutile Ministero per l'attuazione del programma *(Applausi dal Gruppo PD)*, perché in tutti i Paesi democratici

Non ci si dica comunque che non c'erano strade diverse: c'era la strada di istituire il Ministero della salute senza aumentare il numero dei Ministri e dei Sottosegretari. La seconda ragione della nostra opposizione è che questo Ministero nasce con una curiosa subalternità:

nessuno di noi pensa che si possa continuare con la bella vita dello spendere di più, come diceva il collega Cursi -magari nelle Regioni dove si dà di meno in termini di qualità e assistenza - senza che questo comporti (come giustamente fatto dai precedenti Governi e dal ministro Turco) un patto per la salute, impegni assunti dalle Regioni e, se necessari, severi piani di riordino e addirittura commissariamenti. Dunque, sulla necessità del rigore nei conti e di rendere conto di tale rigore non c'è discussione. Tuttavia, che assetto di Governo è quello di un Ministero che per qualunque provvedimento deve prima chiedere il permesso? Il concerto si fa nel Consiglio dei Ministri: se noi conferiamo a questo Ministero una debolezza strutturale nel rapporto con l'Economia, è chiaro che i risultati che ne potremo avere saranno inferiori a quelli auspicabili. Vorrei segnalare a tutti voi colleghi l'intervento molto apprezzabile del collega Rizzi, che peraltro è un operatore operatore della sanità pubblica, il quale ci segnala che quelle esigenze di governo del sistema e anche di una funzione statale sui temi della sanità sono avvertiti da tutte le componenti del Parlamento. Vi segnalo ed è una delle ragioni per le quali il nostro sarà un voto di astensione, che il ruolo che il Ministero dell'economia assume in questa materia può essere in una falsificazione dei dati, e sostanzialmente è sbagliato. I piani di rientro devono essere soltanto di competenza del Ministero dell'economia?

e le stesse scelte di alcune Regioni, in particolare quelle del Mezzogiorno, impegnate nei piani di rientro senza il supporto delle altre Regioni e di un Ministero che funzioni nelle scelte del Governo sulle politiche sanitarie, rischiano di rendere il Ministero della salute, come è stato per molti anni in passato,

proposto dal ministro Sacconi volta a ridimensionare il peso della spesa pubblica del sistema sanitario nei prossimi anni per dare forza a quello che viene definito in quel documento il pilastro privato. Non va bene, perché dove è più forte il pilastro privato lì è più forte, in assenza di regole, di controlli di qualità, di sistemi di verifica e misura, la spesa inappropriata; è più forte la spesa e minore la qualità. Insomma, sulla sanità questo Parlamento dovrebbe tornare a pensare ad una politica che serva al Paese. La terza e ultima considerazione che motiva il nostro voto di astensione

Queste cose si fanno insieme. Le ultime Conferenze Stato-Regioni sono saltate. L'accordo sulla legge finanziaria e sulla definizione dei *budget* per la sanità non ci consente neanche più un dialogo. C'è l'idea di un rapporto di forze per cui il Governo è autosufficiente nella sua maggioranza e va contro tutto; ma si può andare contro tutto? Contro l'opinione delle Regioni e dell'opposizione parlamentare? Quello che mandiamo oggi con un voto di astensione è un segnale alla maggioranza: sulle grandi scelte che riguardano il Paese è necessario, più di quanto non siamo stati tutti noi capaci di fare finora, che si ragioni nel merito e si cerchino le intese. Se questo può avvenire, il voto di astensione che noi diamo è un'apertura ad un ragionamento sul futuro, sulle regole, sul funzionamento di questo Stato, che credo abbia bisogno di una maggiore responsabilità collettiva della sua classe dirigente e politica. Presidente, colleghi, signor Vice Ministro, annunzio il voto convintamente favorevole del Popolo della Libertà su questo provvedimento. Siamo convinti della bontà del medesimo e a questo ci porta una valutazione che aveva trovato nel giugno del 2008 il consenso dell'opposizione.

giorno di maggioranza e di opposizione in relazione al provvedimento di ripacchettamento dei Ministeri, in ossequio all'ultima finanziaria di Prodi, che chiedevano si provvedesse ad istituire il Ministero della salute in modo autonomo e separato rispetto al Ministero del lavoro, della previdenza e della salute. Il Governo disse che avrebbe studiato la situazione, dimostrandosi già allora favorevole attraverso l'accoglimento di quegli ordini del giorno. giorno. Non capisco perché in quest'Aula, oggi, quando si va a realizzare quello sul quale tutti erano d'accordo, ci siano dei Non credo che ciò derivi soltanto dal fisiologico senso di contrasto tra maggioranza e opposizione, ma devo dire che non trovo congrue, non trovo congrue, almeno a mio avviso, le motivazioni sottese alle dichiarazioni di voto.

Vediamo questo Ministero investito dei livelli essenziali, delle prestazioni sociali e civili, competenza pertanto dello Stato, nonché di quella competenza statale anche in materia di legislazione concorrente che tende a determinare i princìpi fondamentali. Sono emersi interventi che ci hanno fatto comprendere come ci sia necessità di un'istituzione centrale che vada a organizzare determinati strumenti

Quando si è allora raggiunta la concreta condivisione su questi argomenti sostanziali, non riesco a comprendere per quale ragione si cerchi di sostenere che l'intervento del Ministero dell'economia finirebbe per snaturare o limitare queste competenze. Abbiamo letto bene quali sono le competenze attribuite dal provvedimento che stiamo per votare? Esse sono le stesse competenze contenute in uno specifico provvedimento precedente,

questa pandemia di influenza) e per far comprendere che è necessaria un'autorità centrale per dare suggerimenti alle Regioni su problematiche complesse di ordine medico.

«per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai Piani di rientro regionale».

Mi pare che non si possa assolutamente sostenere che il Ministero dell'economia vada a cercare competenze ulteriori e in qualche modo non chiare rispetto a questa norma al nostro esame.

riferito all'organizzazione dei servizi sanitari, alle professioni sanitarie, ai concorsi e allo stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, cioè esattamente alle materie già comprese nella legge esistente.

servono dei tempi che, in qualche modo, prescindono dalla necessità di istituire oggi un Ministero della salute. del senatore D'Alia, in qualche modo speculare all'atteggiamento dell'UDC in termini di voto contro il federalismo fiscale (cioè sostenere che l'attribuzione delle competenze sulla salute in via concorrente alle Regioni ha fatto sì che, negli anni, la sanità sia peggiorata), è un'affermazione attinente, comunque, a un'eventuale futuro. non realizzando oggi questa riforma noi ci proietteremmo verso attese future di anni, non andando incontro alle attuali esigenze dei cittadini.

e danno 500 milioni di euro ai loro amici e sodali come Zunino (Risanamento S.p.A.), seppellito sotto 3 miliardi di euro di buco. Il sistema bancario ha la complicità collusiva della Banca d'Italia che, invece di vigilare sulla correttezza e trasparenza, va a braccetto con i banchieri. Se una famiglia colpita dalla crisi non riesce a pagare il proprio mutuo perde la casa costata sudore e sacrifici; se le banche, dopo aver praticato l'usura legalizzata denominata anatocismo, vengono condannate dai tribunali a risarcire l'illecito si permettono di non ottemperare alle sentenze esecutive e a non pagare. È accaduto in questi giorni al tribunale di Lanciano: per una sentenza esecutiva, solo

Mi permetto ancora una volta di richiamare l'attenzione del Governo sulla protezione della Banca d'Italia, che non deve vigilare solo sulla stabilità del sistema, ma anche su comportamenti illegali e che è obbligata a

questo Governo non fa nulla per arginare lo strapotere del sistema bancario e la vergognosa collusione della Banca d'Italia, che non fa nulla per ripristinare la legalità bancaria. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo e del Ministro dell'economia, sollecitati da numerose interrogazioni e

non può essere più consentita. Questa Banca d'Italia non può più continuare a lavarsene le mani. Si dice che il Super Mario de' noantri, Mario Draghi, lo mandiamo in Europa: dopo aver fatto danni all'Italia

rispetto ad un'interrogazione che pure riguarda un tema molto importante che credo stia molto a cuore a questo Governo: il tema dell'informazione e, in particolare, di quella locale.

televisive locali che, per essere delle televisioni commerciali, si sentono *legibus solutae* e quindi, come tali, disponibili a fare e a dire di tutto di più per il solo fatto che a volte trovano qualche Corecom compiacente. Il più delle volte, grazie a questa compiacenza, riescono ad avere l'erogazione di somme notevolissime che coprono quelle che sono evasioni di carattere fiscale e contributivo, il che naturalmente le legittima a fare di tutto di più in assenza di un intervento del Governo.

andassero a emittenti locali pugliesi che non hanno assolutamente i requisiti per poter accedere ai contributi. Non si può chiedere, da un lato, agli italiani di stringere la cinghia e, dall'altro, agevolare l'evasione e l'illegalità da parte di un sistema televisivo locale che il più delle volte procura danni notevolissimi piuttosto che dare un'informazione corretta.

presenti ad Aversa, si è incancrenita una situazione di disagio per tutti gli utenti, malgrado i centri vicini, in modo particolare la città capoluogo, abbiano più del doppio degli uffici postali.